Grazie a tutti la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 624. **Sull'ordine

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine del giorno per comunicare, ritenendolo utile per il dibattito dell'Assemblea, che l'Ufficio di Presidenza della 6a Commissione, nella seduta di ieri, ha deliberato la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione della crisi e la garanzia dei depositi europei. Questa indagine conoscitiva è stata avviata nel febbraio 2016 e ha svolto 23 audizioni che hanno visto impegnati esponenti del consiglio di vigilanza della BCE, della magistratura, della Banca d'Italia e di associazioni di categoria. L'indagine conoscitiva veniva considerata prodromica alla Commissione d'inchiesta auspicata in più disegni di legge. Come dicevo, ieri l'Ufficio di Presidenza, anche alla luce del dibattito che si era sviluppato sia in Aula sia sui *media*, ha ritenuto che non fosse opportuno restringere il campo dell'azione svolta

era stato fatto con lo spirito di rendere subito operativa quella ricerca di trasparenza che ritenevamo necessaria per un tema così delicato. Come dicevo, quindi, l'Ufficio ne ha deliberato la conclusione, stabilendo il deposito della relazione conclusiva per il 17 gennaio, la votazione della stessa per il 25 gennaio e l'avvio della procedura legislativa per la Commissione d'inchiesta in 6a Commissione il 31 gennaio

Come dicevo, la volontà di poterci occupare di tutto questo, continuando un'azione che è stata svolta proficuamente con la collaborazione di tutti i commissari, ci ha portato a questa risoluzione. Volevo comunicare all'Assemblea queste determinazioni sperando che potessero costituire un elemento utile per il dibattito. *(Applausi

Signor Presidente, mi faccia preliminarmente esprimere i miei auguri di pronta guarigione al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni

comE è logico e come prevedono i nostri Regolamenti. Abbiamo sentito poco fa che la Commissione finanze, dopo una seria e necessaria indagine,

Oggi, però, noi siamo chiamati ad esprimerci sull'urgenza, di fatto superata dalla decisione della Commissione finanze, di un solo disegno di legge che rappresenta soltanto una parte delle iniziative legislative all'esame del Senato.

riguardi un solo disegno di legge, ma l'insieme di quelli oggi all'esame della Commissione finanze, che, come abbiamo sentito, sono tutti egualmente urgenti.

La nostra priorità assoluta è la piena trasparenza. Questo è l'obiettivo ed è la prima ragione per la quale i senatori del Gruppo del Partito Democratico hanno presentato tra i primi, più di un anno fa, una proposta di Commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Chiediamo, quindi, trasparenza e non altro. Il Parlamento e gli italiani debbono sapere perché alcune nostre banche sono andate in crisi e comprendere quali rimedi vengono approntati. Abbiamo anche un profondo rispetto per il sistema bancario italiano, di cui conosciamo la complessiva condizione positiva e del quale ben conosciamo il delicatissimo ruolo per la nostra economia e stabilità e anche per la stessa nostra sicurezza nazionale, che proprio in queste ore vediamo seriamente insidiata su altri e altrettanto delicati comparti. In tempi così difficili come i nostri, Presidente, la Commissione d'inchiesta dovrà, quindi, trovare una strada anche normativa per raggiungere il massimo risultato in termini di trasparenza, mantenendo intatta la forza, la credibilità e il prestigio del nostro sistema bancario.

consente a questa Camera di parlare della Commissione d'inchiesta; ma la Camera ieri ha approvato all'unanimità, su proposta dell'omologo di Forza Italia, presidente Brunetta, una mozione - leggo testualmente la parte finale del dispositivo - che «impegna se stessa, i propri organi, ciascuno per le proprie competenze, a deliberare in ordine all'istituzione di un Commissione parlamentare d'inchiesta

nell'evoluzione che ha subito e nelle parti che hanno rappresentato un problema per i risparmiatori che hanno investito. Siamo d'accordo anche noi che la procedura di urgenza, a questo punto dei lavori del Senato, riguardi tutte le iniziative legislative che potrebbero determinare alla fine la

le due Camere a decidere quale sia il percorso iniziale che dovrà essere fatto. Dico solamente e sommessamente che, visto che in questa sede abbiamo il provvedimento sul e il milleproroghe, nel bilancio complessivo potrebbe essere corretto che sia la Camera ad affrontare in prima lettura il disegno di legge di istituzione della Commissione d'inchiesta, altrimenti andremmo ad affollare questo ramo del Parlamento a discapito dell'altro. Comunque è un problema di

però, significa tempi dimezzati, lo sappiamo benissimo; altrimenti è inutile che deliberiamo l'urgenza. Alla Camera è stata approvata una mozione per impegnare la Camera Sappiamo benissimo - e lo abbiamo già visto con la pubblicità sul gioco d'azzardo - che, quando le due Camere sono impegnate sullo stesso argomento quando c'è l'urgenza sul medesimo argomento nei due rami del Parlamento, si blocca tutto. Non vorrei quindi che questo fosse un giochino per poi rallentare l'effettiva costituzione della Commissione d'inchiesta. In Ufficio di Presidenza abbiamo deliberato che, se non ci fosse stata l'urgenza, saremmo partiti il 31 gennaio.

è il solito lancio della notizia che la maggioranza in qualche modo è d'accordo a difendere i cittadini italiani, ma poi tutto si blocca. Noi siamo dunque favorevoli

Signor Presidente, naturalmente anche il Gruppo della Lega Nord è favorevole ad affrontare il tema della Commissione d'inchiesta nella sua complessità e non solo relativamente alla situazione del Monte dei Paschi, che forse è la più grave, ma non è l'unico problema del mondo bancario italiano. È giusto fare una riflessione complessiva, però vorrei anche dire al Presidente del Gruppo del Partito Democratico che qui non è il Partito Democratico che accelera, perché il Partito Democratico per un anno ha tenuto fermo in Commissione finanze l'*iter* per l'approvazione di questa Commissione d'inchiesta. È passato più di un anno dal novembre 2015, quando sono state depositate le proposte di legge. Noi, da subito, in Commissione finanze abbiamo dichiarato che era inutile fare un'operazione conoscitiva, con 23 audizioni, per varare questo tipo di Commissione d'inchiesta, perché era già stata fatta. Si è trattato di un'inutile ripetizione, attuata consapevolmente dal Partito Democratico con un solo intento, dilatorio e di rinvio, per non affrontare questa delicata tematica. Abbiamo perso più di un anno per vostra responsabilità. Ora c'è un'improvvisa accelerazione da parte vostra, dopo la riunione Democratico al Nazareno. Ma, onestamente, che si venga a dire che il Partito Democratico è determinato ad andare in questa direzione, che vuole accelerare e che non teme la trasparenza contrasta con quella che è stata la realtà dei fatti negli ultimi tredici mesi, mesi di inattività, di inerzia e di colpevoli ritardi, durante i quali la situazione del mondo bancario non è migliorata, ma è addirittura peggiorata. peggiorata. Quindi, basta colpevoli ritardi; sicuramente bisogna accelerare. A questo punto chiediamo certezze anche perché siamo evidentemente a fine legislatura e probabilmente siamo anche oltre tempo massimo. Faccio un'ultima osservazione: noi riteniamo che, dopo per un anno si è affrontato questo tema in Commissione finanze, con tutta una serie di audizioni, il luogo deputato ad avviare l'*iter* per l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta debba essere il Senato, a meno che quel lavoro venga messo a frutto e non sia gettato al vento con un *iter* che dovrà ricominciare alla Camera dei deputati. Concludo il mio intervento confidando confidando che questa attuazione venga portata avanti in un modo accelerato, così come richiesto anche dalla collega del Movimento 5 Stelle, senza inutili, ulteriori ritardi.

citare i casi più significativi: dalla banca delle Marche alla Banca popolare dell'Etruria, alla Cassa di risparmio di Ferrara a quella di Chieti; Banca popolare di Vicenza, Banco di Desio e della Brianza, Veneto Banca.

- oggi il Senato assumerà con il voto, arriva con un certo ritardo. Lo voglio sottolineare perché anche ieri, durante la discussione in Commissione affari costituzionali sul decreto-legge salva banche, abbiamo fatto presente che per un lungo periodo

Per quanto riguarda la questione della

diceva Bauman, scomparso proprio qualche giorno fa, che il più grande ostacolo a trovare risposte è la nostra lentezza nel cercarle. È innegabile che su questo tema qualche lentezza l'abbiamo accumulata. Certo, la complessità e la delicatezza del tema e del suo sistema, interessato

ancora una volta, di trattare il tema con l'urgenza, la cautela e la responsabilità che questo caso, come altri, merita. Noi dobbiamo però ricordare che il percorso che ci ha portato stamane qui in Assemblea si ripete per la seconda volta, dopo che qualche mese fa io a chiedere, con la procedura d'urgenza, di poter valutare se fosse giunto e fosse ormai maturo il tempo per consentire al Parlamento di riappropriarsi di un ruolo che non è quello delle inchieste

delle vigilanze e delle burocrazie italiane ed europee nell'affrontare correttamente quel problema che oggi vediamo sulle spalle dei risparmiatori in virtù di un *bail in,* che quest'Assemblea ha votato con grande leggerezza.

affrontare il doloroso tema del *bail in* ed essere pronti, con un decreto-legge che quest'Assemblea esaminerà per prima, a mettere in moto il meccanismo del *bail out*.

che rischia di sconquassare il sistema economico, se non anche la tenuta sociale di alcuni territori. L'oggetto della Commissione d'inchiesta oltre alla trasparenza che è il primo obbligo che abbiamo verso il cittadino, il quale non è sempre nelle condizioni di poter comprendere appieno ciò che legge sui giornali o le informazioni che riceve. Del resto, come poteva farlo quel cittadino quando in tanti anni di pensiero unico sulla finanza ingegnerizzata e degenerata si sono lette intere pagine di assoluta adesione a un modello finanziario tanto diverso dal nostro da aver creato sconquasso nel mondo e oggi nel nostro Paese aver minato profondamente la tenuta di quel risparmio

lavorato su questo fronte da tempo intraprendendo, attraverso l'indagine conoscitiva, un preciso e profondo lavoro di raccolta di informazioni che oggi costituiscono il miglior substrato per poter valutare in una Commissione d'inchiesta quali sono i confini di questa inchiesta e cosa ci interessa davvero far emergere in essa. A me interessa che il Parlamento sia pienamente consapevole di ciò che è accaduto di ciò che è accaduto sul piano della proposta del credito nel nostro Paese, che non è solo il frutto di una crisi partita nel 2008 attraverso sistemi finanziari tutti ispirati a una logica di profitto rapido e immediato che hanno determinato uno *shock* finanziario

Per questo ringrazio tutti i colleghi della Commissione che hanno fatto, come me e molto meglio di me, un lavoro certosino e preciso che oggi è il miglior modo per essere rapidi. Per essere rapidi sul serio e concreti occorre partire da lì, proseguire su quella strada e rendere il più presto possibile all'Assemblea un prezioso lavoro di conoscenza e di consapevolezza di qual è la vera posta in gioco, che è il ruolo di questo Parlamento e non il sostituirsi ad altri poteri e ad altre responsabilità. La nostra responsabilità è invece quella di sapere, conoscere e legiferare su un tema che ci riporta indietro di tanti anni, per poter mettere in evidenza come una grande legge bancaria dopo la crisi del 1929 aveva tenuto il sistema economico nel suo insieme, soprattutto quello europeo e quello occidentale, in un grande equilibrio

A noi interessa la trasparenza totale su quanto accaduto. A noi interessano la conoscenza precisa di tutti i meccanismi e anche le ipotesi di modifiche legislative, che possano mettere in grande solidità il nostro sistema bancario. Ci interessa questa solidità bancaria, perché abbiamo un senso di grande responsabilità verso i nostri cittadini e perché dobbiamo tutelare i nostri cittadini che certamente sono, in questo momento, assolutamente sbandati, senza alcun tipo di certezza rispetto a una situazione che riguarda non solo la banca sulla quale stiamo facendo un ragionamento preciso e puntuale con un decreto, ma tutto il sistema bancario nazionale. Per questo anche noi, signor chiediamo che la Commissione d'inchiesta possa analizzare i tredici disegni di legge depositati in Commissione,

oggi stanno indagando su questo caso. Noi siamo il Parlamento e dobbiamo dare solidità. Noi dobbiamo conoscere e garantire trasparenza. Noi dobbiamo tutelare i nostri cittadini

la questione sta nei seguenti termini. Questo disegno di legge avrebbe bisogno di andare avanti da solo,

per il volume di denaro che coinvolge, per i problemi che ha creato e per la durata della situazione. Il Monte dei Paschi vale dieci volte

Ho chiesto di intervenire dopo l'intervento del senatore Santangelo per sostenere che quella tesi era corretta e lei non mi ha dato la parola.

Ne prendo atto. L'Aula si è pronunciata e anche il suo Gruppo è intervenuto. Noi abbiamo applicato l'articolo 92 del Regolamento. Tutti i Gruppi si sono pronunciati e poi abbiamo votato.

È incredibile, perché l'articolo 92 non recita assolutamente quello che lei ha detto. La invito a leggerlo all'Assemblea, perché è impossibile che il Senato possa essere guidato con questa modalità. Questa volta il senatore Zanda ha fatta una richiesta, ma la richiesta del senatore Zanda ha motivo di esistere ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento: la richiesta avanzata dal senatore Zanda non può assolutamente essere accorpata con la richiesta fatta in precedenza, signor Presidente,

al disegno di legge n. 624. La Presidenza ritiene quindi assorbita la questione dell'articolo 77 dal voto precedente, sul quale - le ribadisco - i Gruppi hanno avuto possibilità di esprimersi ai sensi del Regolamento: anche il suo Gruppo si è espresso a favore.

un momento la parola per riprendere il percorso dal punto in cui l'avevamo lasciato, perché molti ricordano che erano stati espressi i pareri sugli emendamenti,

Ricordo di aver formulato l'invito agli estensori degli emendamenti 8.201 e 8.203 (l'emendamento 8.202 era stato ritirato) a convergere sull'emendamento 8.206,

ed è un modo molto efficace per raggiungere una conciliazione o anche una proposta effettiva di mediazione e di transazione sul procedimento. Prevedere la media conciliazione significa

perché spesso sono praticamente inutili. Se la media conciliazione non la si fa con una perizia, praticamente l'attività svolta, che il cittadino deve pagare, perché la media conciliazione va pagata, Parimenti, anche se non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, è ovvio che se si fa un tentativo di conciliazione con un'azienda ospedaliera e con medici per casi di responsabilità sanitaria, che tra l'altro sono molto complessi, è impossibile farlo da solo,

l'emendamento 9.218 è molto semplice e permette di specificare il momento di riferimento per la quantificazione del massimale poiché dette norme, nell'attuale formulazione, lasciano incertezza in merito alla determinazione del massimale stesso. Grazie

dell'ospedale di Nola che abbiamo visto in questi giorni e che hanno fatto riscontro ad una serie numerosa di dichiarazioni, alcune veramente improvvide e incredibili nel loro contenuto, mi aiutano e mi sorreggono nel motivare la presentazione dell'emendamento 10.201. Le attuali polizze assicurative coprono, com'è ben noto, soltanto la responsabilità professionale del medico o, più in generale, del personale sanitario per motivi di negligenza, di imprudenza e imperizia. Non è previsto che venga estesa la copertura anche ai casi in cui il danno sia determinato dal *deficit* strutturale cagionato da negligenze da parte dell'amministrazione.

danno che eventualmente il paziente potrebbe ricevere non essendo ricoverato in un letto ma depositato - oserei dire - a terra non può ricadere sul medico o sul personale sanitario: evidentemente deve ricadere su su una amministrazione negligente che non è stata capace di realizzare le strutture idonee. anche per motivi inerenti a *deficit* strutturali e organizzativi rispetto ai quali gli operatori della sanità non hanno di fatto un livello di corresponsabilità, ho pensato di proporre, attingendo al patrimonio di buonsenso, questo emendamento che prevede che venga introdotta la previsione che i danni possano essere cagionati non soltanto per responsabilità professionale del medico e del personale sanitario, ma anche da carenze strutturali e organizzative di presidi, determinati dalla carenza di organico, che sono evidentemente imputabili alla gestione dell'ente. dell'ente. Credo si tratti di un emendamento che possa essere accolto e, in tal senso, formulo il mio auspicio.

visto che tutte le strutture sanitarie hanno dei uffici legali, che siano questi a scegliere e a chiedere all'assicurazione che assicura la struttura di predisporre delle polizze per i professionisti sanitari (che loro stessi pagheranno).

Grazie

Grazie

Con l'impianto previsto da questa nuova normativa si prevede espressamente un'azione diretta da parte del danneggiato nei confronti del medico.

signori, che medici che esercitano professioni quali quella del ginecologo (in materia proprio di ostetricia) o del neurochirurgo hanno dei preventivi per polizze assicurative che superano i 10.000 o i 15.000 euro annuali. Si sta parlando di somme che sono inaffrontabili da parte di medici attualmente incardinati all'interno di strutture ospedaliere, i quali possono vantare delle retribuzioni che non gli permettono sicuramente di affrontare questi carichi. Noi abbiamo sollevato questa problematica riguardo a questo disegno di legge.

e delle ASL. Il singolo che si trova ad affrontare il mondo del mercato delle compagnie assicuratrici non ha la possibilità e la capacità (con tutto il rispetto, perché ognuno fa il suo lavoro) di scegliere quale sia la polizza più adeguata.

che permetta di avere il premio più basso, perché a volte il premio basso è associato a condizioni che magari non coprono tutto. Vi porto l'esempio di quanto è stato fatto dalla Regione Veneto. La Regione Veneto si è resa conto di questa difficoltà

Con questo non si deve intendere che le ASL stipulino polizze a favore dei dipendenti, come abbiamo anche proposto, perché comprendiamo quali possono essere le difficoltà normative.

un mondo veramente molto difficile. Per cui noi, con questo emendamento, continuiamo ad insistere su questa problematica. Ben venga venga una ristrutturazione, una revisione di tutto l'ambito della responsabilità medica sotto il profilo giuridico, che è comunque complesso, ma dobbiamo tener conto della parte assicurativa.

riguarda l'obbligo di assicurazione. Nell'articolo 10 diciamo infatti che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa; quindi, c'è un'obbligatorietà per queste strutture di dotarsi di copertura assicurativa. L'emendamento che ho presentato, il 10.203, estende l'obbligo di contrarre alle imprese assicuratrici perché

che le assicurazioni non stipulino polizze alle aziende sanitarie pubbliche e private. Se parliamo in particolare delle aziende pubbliche, per poter contrarre una polizza un'azienda pubblica deve fare una procedura a evidenza pubblica: non può stabilire una contrattazione di tipo privato o una trattativa privata plurima con più soggetti assicurativi; deve indire una gara di appalto, che ha i suoi tempi e costi, e soprattutto deve stabilire parametri precisi per poter preparare un capitolato d'appalto. Se a questa gara, per esempio, non partecipa nessuno perché non c'è alcun obbligo di nessun genere, come farà mai un'azienda sanitaria a dotarsi di una polizza assicurativa?

si pensa di rimandare il tema alla discussione che faremo sul decreto-legge concorrenza, il quale probabilmente conterrà norme che riguarderanno le imprese assicuratrici;

10. Pensate per un attimo alle immagini che stanno facendo il giro d'Italia dal punto di vista mediatico, che riguardano l'ospedale di Nola, vicenda che si arricchisce ogni giorno di nuovi spunti e nuovi elementi. se pensiamo a quello che è successo in quell'ospedale (dove la responsabilità dei medici emerge a fronte di una carenza d'informazione presunta rispetto all'azienda sanitaria locale e quindi alla direzione generale),

Grazie sia pubbliche che private potrebbero non avere la possibilità di contrarre alcuna polizza, quindi questo articolo sarebbe vanificato e resterebbe inattuato proprio per la difficoltà, o meglio per la mancata volontà

che - vi chiedo di fare attenzione - inviti il Governo a valutare le modalità attraverso le quali le Regioni (qui dobbiamo metterci d'accordo, se le Regioni o le aziende, che sono due cose diverse)

un ordine del giorno che esorti il Governo a valutare le modalità attraverso le quali i professionisti possano accedere a

in altri provvedimenti), potremmo creare le condizioni per cui i direttori generali o anche gli stessi responsabili medici, non avendo polizza assicurativa, siano portati a violare un articolo di legge che stiamo approvando questa mattina.

che probabilmente ha poca conoscenza di un contratto. Dire che già nella norma licenziata dalla Commissione è prevista tale possibilità è del tutto sbagliato, perché quando si stipula una polizza di assicurazione e vi è l'obbligatorietà di tale polizza assicurativa

Grazie a tutti il rapporto contrattuale è governato dall'autonomia negoziale: mentre noi possiamo imporre alle strutture pubbliche di munirsi di una polizza assicurativa, non possiamo imporre a un soggetto privato una determinata attività è questa la ragione. Per quanto io apprezzi il senso e le finalità dell'emendamento, c'è questa forzatura che da

che era di buon senso, ragionevole e che comunque era opportuno fosse inserito nella norma proprio per le ragioni che ho detto. Infatti, prevedere la stipulazione e la obbligatorietà di una polizza senza contenuti non ha senso.

da diverse spese di assistenza per i cittadini. Non forniamo, cioè, le siringhe agli ospedali e con quei soldi imponiamo all'ente di stipulare una polizza inutile, che non serve a niente, perché non si sa cosa andrà a coprire. Se questo è un modo di governare la sanità nel nostro Paese, allora io devo dissentire, da cittadino prima ancora che da parlamentare. Non è sopportabile, peraltro, quella arroganza. Tutti ormai hanno parlato di Nola. Ebbene, io sono anche stanco, perché le dichiarazioni e i provvedimenti assunti dal Governatore della come la sospensione del direttore sanitario e di altri sanitari di quella struttura, non meritano neanche di essere commentati, in quanto espressione di una arroganza, di una scostumatezza istituzionale, di una incompetenza, di una incapacità e di di una incapacità e di un atteggiamento fascista, ma non di quei valori portati dagli amici dell'allora Movimento sociale italiano, bensì di quei valori più beceri che la storia ha del senatore Barani).* Noi oggi abbiamo ancora qualche espressione di tal genere tra coloro che amministrano le nostre strutture e i nostri organismi. E ahimè, lo dico da povero cittadino campano, proprio la mia Regione è governata in questo modo.

sempre di più alla possibilità che, se si verifica un fatto rilevante come quello di una invalidità permanente o di un danno letale, ci ritroviamo con un'accusa perpetrata nei confronti del sistemo medico e sanitario, Grazie a tutti la categoria sanitaria, in presenza inoltre di un sistema assicurativo, quello italiano, parzialmente inadeguato (bene ha fatto il collega Cuomo a evidenziarlo con il suo emendamento)

imporre dal punto di vista pubblico che le compagnie assicurative italiane debbano andare a offrire una garanzia di responsabilità civile e professionale al committente e al richiedente; evidentemente, però, ciascuna compagnia che non intenda assumere quel rischio ha un margine di possibilità operativa nel non offrire una tariffa adeguata alle condizioni economiche del richiedente, ponendosi così al di fuori delle disponibilità. Quindi, offrire un'opportunità di copertura assicurativa non significa automaticamente poterla stipulare,

Il problema resta. Siamo in quella terra di mezzo in cui non esistono ancora compagnie molto specializzate nel settore della responsabilità civile professionale adeguate ad offrire tariffe di mercato ma, nel contempo, ad avere quella capacità di analisi, anche finanziaria ed economica, che permetta loro di offrire una copertura in cambio di un premio, ovvero di una tariffa adeguata. Il problema posto dal collega Cuomo è tutt'altro che irrilevante e non lo vedo completamente risolto dal disegno di legge in corso.

possano effettivamente trovare sia sul mercato assicurativo sia dal punto di vista della premialità, quindi del costo assicurativo, un'adeguata risposta nel mercato italiano.

norma molto combattuta dalle compagnie assicurative, che fu introdotta nell'ordinamento italiano all'interno del testo unico sulle assicurazioni private e che fu attaccata proprio dalle compagnie assicurative. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare ancora una volta un regalo alle compagnie assicurative non inserendo l'obbligo a contrarre anche per queste fattispecie di assicurazione professionale sanitaria? In un certo qual senso, se non si inserisce l'obbligo a contrarre noi diamo ancora una volta il coltello dalla parte del manico alle imprese assicurative.

ne parlò in maniera molto favorevole dicendo che si trattava di una norma a favore dei cittadini, cioè a favore della controparte nel contratto assicurativo. In questo caso la controparte rispetto alle compagnie assicurative sono gli enti pubblici sanitari. Quindi noi cosa vogliamo fare? Ancora una volta non abbiamo fatto esperienza?

e dando tale possibilità - come l'abbiamo data allora ai cittadini, controparti delle compagnie assicurative - ai nostri enti pubblici, che diventeranno controparte rispetto alle compagnie assicurative.

ascoltato la puntuale ed ampia valutazione e illustrazione che il collega Cuomo ha fatto del suo emendamento, e illustrazioni che i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto per meglio comprendere il punto di criticità che si intende affrontare.

di un impegno al Governo ad affrontare quello che può essere un punto di criticità. Dobbiamo assolutamente evitare il rischio che la mancata approvazione di questo emendamento possa determinare un *vulnus* nell'ambito dell'approvazione del disegno

vorrei soltanto segnalare che questo provvedimento è stato lungamente esaminato, per più di un anno ormai, dalla Commissione sanità ed è stato esaminato in prima lettura dalla Camera Il punto in discussione nasce da un'esperienza concreta. Dobbiamo sapere che negli anni passati le imprese assicurative non avevano più alcuna intenzione di assicurare il punto delicato su cui abbiamo cercato di lavorare è quello di contemperare le esigenze del mondo sanitario con l'impossibilità, perché sarebbe patetico, di condurre e dirigere un mercato, come quello assicurativo, attraverso un provvedimento di tipo sanitario. È chiaro che l'argomento si completerà la legge sulla concorrenza, che è la sede propria in cui discutere di questo argomento, e non inserendo una parte che sarebbe sinceramente

come abbiamo detto più volte, come il relatore ha espresso nella sua relazione e il dibattito che si è svolto fuori di qui ha rimarcato più volte. È un tema che va però inserito nell'ambito corretto che è quello della concorrenza, anche perché vi sono elementi tecnici che possono essere definiti solo da una legge di quella natura. Per cui ritengo che la presentazione di un ordine del giorno possa contemperare le esigenze che sono state sollevate da diversi colleghi con colleghi con l'esigenza però di mantenere un testo che è già molto complicato e dettagliato nei termini che la materia richiede.

ma anche e soprattutto per le aziende sanitarie ed i pazienti, i quali avrebbero maggiore certezza di ottenere le somme rispettivamente riconosciute alle prime in sede di rivalsa ed ai secondi a titolo di risarcimento del danno. Si precisa inoltre che questa norma, così come è formulata, risulta conforme alle disposizioni inerenti alle coperture assicurative delle altre professioni, quale ad esempio il decreto del Ministero di giustizia del 22 settembre 2016, che disciplina le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative per gli avvocati.

Quando viene denunciato un sinistro, considerando che nei casi di responsabilità medica vi può essere la previsione di somme ingenti a titolo di risarcimento del danno, spesso l'assicurazione presenta poi la disdetta ai sensi del contratto. Ovviamente, questo crea problematiche non da poco. Per questo abbiamo ritenuto di inserire la previsione per cui nelle condizioni di polizza dev'essere previsto obbligatoriamente il divieto di recedere da parte dell'assicuratore nel caso di una denuncia di sinistro.

in cui è stato asserito che non si poteva prevedere un obbligo per le assicurazioni di contrarre polizze, non capisco per quale motivo possiamo invece prevedere un obbligo per le assicurazioni di estendere la garanzia assicurativa. Se non possiamo prevedere un obbligo in un modo, non vedo per quale motivo potremmo poi prevederne un altro. Voler spostare i riferimenti normativi che ci impegnano su questo disegno di legge ad un successivo provvedimento sono abbastanza inusuali per un'Assemblea parlamentare e per questo motivo,

di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Ecco, questo è un comma di cui chiedo la soppressione, in quanto spinge i professionisti sanitari ad una medicina di tipo astensionistico,

Presidente, come Gruppo della Lega Nord abbiamo proposto emendamenti volti sia a sopprimere il comma 3, sia eventualmente a formularlo in una maniera diversa al fine di evitare proprio ciò che veniva anticipato. Quello che si vorrebbe assolutamente evitare che il medico si trovi nella difficoltà di temere l'azione di rivalsa e in tal senso condizioni il proprio operato al fine di evitare di subire una causa futura. Per questo si parla di medicina astensionistica o addirittura difensiva: nel momento in cui il medico si trova di fronte ad un caso particolare, ovviamente prescriverà l'esame in più, effettuerà magari una TAC in più una TAC in più o troverà l'occasione di evitare di affrontare quella problematica, passandola ad un collega o ad un'altra situazione, proprio per non esporsi.

Noi riteniamo che debba essere inserita nella norma la possibilità che tale fondo intervenga anche nell'ipotesi in cui non vi sia una copertura assicurativa, nel caso in cui l'assicurazione abbia formulato un recesso oppure per difficoltà inerenti la compagnia stessa.

Senatore Bianco, opportunamente sottolinea l'opportunità di individuare un cosiddetto Fondo di Area terapeutica. Il problema nell'ordine del giorno è che tecnicamente le risorse con cui finanziare questo Fondo, che derivano dal fondo di garanzia, sono assolutamente irrisorie. Il merito è corretto, ma la previsione tecnica dell'ordine del giorno

una dichiarazione di voto molto semplice, che parte, intanto, dal metodo seguito. la Commissione sanità abbia dato prova di una politica dialogante che, pur mantenendo ferme le posizioni rinvenibili dalle diverse sensibilità politiche, riesce a trovare punti di equilibrio che vanno nella direzione di intercettare

Sì, *vulnus*, perché di questo bisogna parlare quando si fa riferimento al tema complesso e delicato della responsabilità professionale in ambito sanitario, perché le implicazioni relative all'argomento non sono soltanto quelle più percepite, visibili, conosciute ed emergenti che riguardano la tutela della salute, ma sono anche di natura economica, etica, culturale e addirittura di natura antropologica. Il tema non è nuovo, è antichissimo. Lo scriveva Ippocrate, dicendo: «Che ci siano tra i malati curati dai medici, alcuni che guariscono perfettamente è un fatto che tutti riconoscono; ma siccome non tutti guariscono, per questa ragione l'Arte è ormai biasimata, e quelli che ne dicono male, prendendo a pretesto i malati che soccombono alle malattie, sostengono che chi ne scampa lo deve al caso e non all'Arte».

il rischio che il paziente rimanesse privo di una risposta inerente alla qualità delle prestazioni ricevute e la garanzia che esse fossero

ma più in generale della comunità) oggi trova riscontro e una risposta adeguata. di legge in esame è di iniziativa parlamentare: il mio collega Fucci, membro della Camera dei deputati, è stato il primo firmatario di un disegno di legge avente ad oggetto questa materia. colma un *vulnus* e risolve uno squilibrio nel rapporto tra operatore sanitario e paziente: rivaluta e pacifica questo rapporto attraverso la restituzione dell'atto medico a una dimensione di trasparenza e possibilità di accesso a tutte le implicazioni che, intorno ad esso, si vanno a determinare, restituendo al cittadino diritti che che sino a oggi erano negati. Attraverso questo provvedimento riusciamo a dare maggiore sicurezza alle cure e i principi che ruotano intorno alla gestione del rischio clinico e della prevenzione hanno un riscontro prioritario e rappresentano la stella polare del provvedimento. Ricordo altresì l'obiettivo di una virtuosa circolazione delle informazioni fra i vari livelli istituzionali, da quello centrale e ministeriale, al coinvolgimento dell'Agenas, fino ad arrivare alla struttura sanitaria territoriale. alle linee guida, che rappresentano sostanzialmente le buone pratiche clinico-assistenziali alle quali ci si deve adeguare e alle quali bisogna dimostrare di essersi adeguati,

assolutamente ingiustificato, come ingiustificata era la preclusione del cittadino all'accesso alle informazioni che riguardavano le Un altro aspetto importante è che la medicina difensiva riduce il suo livello di virulenza di virulenza - oserei dire - atteso il fatto che, individuate delle norme che riequilibrano il sistema, indubbiamente non vi sarà più il ricorso a quegli atteggiamenti che nel loro complesso hanno hanno portato a definire medicina difensiva il sistema di protezione che si era determinato per la tutela anche della posizione dell'operatore della sanità. Vi è poi l'effetto deflattivo del contenzioso: sono particolarmente contento del fatto che sia stato accolto un mio emendamento attinente alla possibilità della effetti sui costi delle polizze assicurative, il recupero di vitalità - fatto non marginale - per le scuole di specializzazione che avevano conosciuto il rischio di spegnersi: mi riferisco soprattutto alla ginecologia, all'ortopedia e alla chirurgia, stante la ormai assoluta indisponibilità dei medici a seguire quei percorsi specialistici che erano e sono tra i più alti in termini di conflitto fra medico e paziente. È quindi un aspetto fondamentale che riguarda i profili di tutela della salute, che conferisce alla nostra sanità un livello di qualità certamente superiore, ma che determina anche cospicuo risparmio, se è vero (come è vero)

ammontano i costi del contenzioso medico-legale, che ogni anno registra 30.000 richieste di risarcimento danni per presunte *malpractice*. Io credo che oggi stiamo per

può consegnare al Paese provvedimenti importanti e di questo voglio ringraziare tutta l'Assemblea, tutti i colleghi della Commissione, il relatore il relatore e i colleghi che, con spirito di maturità e con grande senso di responsabilità, hanno contribuito ad animare un dibattito qualitativamente elevato, il cui risultato è scritto nelle buone pagine del provvedimento che andremo ad approvare e che noi Conservatori e Riformisti approveremo con soddisfazione.

Questo provvedimento è stato affidato alla Commissione sanità. Senza nulla togliere alla competenza e al valore dei commissari della 12a Commissione permanente, non ci si può non accorgere che il provvedimento parla squisitamente in termini strettamente giuridici.

Si è parlato per anni del contratto sociale, si è parlato per anni della responsabilità contrattuale, con un insieme di requisiti e di presupposti di azione.

che in parte, tra l'altro, è stato anche recepito, ma la materia doveva essere trattata unitariamente. Ma passiamo al contenuto del disegno di legge.

e paziente è informato necessariamente su un rapporto di fiducia, ed è in quel rapporto di fiducia che risalta la nobiltà dell'attività del medico. Non è vero che il paziente che può denunciare in misura maggiore il medico sarà un paziente più tutelato. L'approccio del medico in questa maniera potrebbe essere influenzato

l'impianto normativo doveva semplicemente prevedere percorsi sanitari, magari con procedure più snelle, in un'ottica di totale collaborazione e ribaltando quell'idea per cui l'indennizzo e il risarcimento sono sinonimo di fallimento o di imperdonabile errore medico. Signori, la medicina, propriamente, non è una scienza, ma un'arte.

Per aiutarmi in questa dichiarazione di voto, perdonatemi se faccio ora mie parole che non sono sicuramente di un avvocato o di un parlamentare, ma di medici.

Sono anni che raccontano che medico e paziente sono ormai diventati le controparti; che il paziente, per essere tutelato, deve poter denunciare il medico; e che il medico, per ben curare, deve avere sul collo il fiato di avvocati, assicuratori e giudici. E così E così il medico, per proteggersi, è bene che scriva sempre tutto, anche le cose più banali e inutili. Più scrivi e più ti autotuteli. Cartelle cliniche ormai diventate dei tomi enciclopedici, consensi informati ormai sovrapponibili a contratti di acquisto; descrizioni di atti operatori simili a compendi di anatomia, di fisiologia e di tecnica chirurgica, intramezzati da commenti quali «non essendo possibile», «vista la situazione», «in considerazione del quadro», «alla luce del referto intraoperatorio». Quasi tutto fosse già pronto e destinato a un dibattito processuale. Dietro a tutto ciò, che non è comico considerata la drammaticità dell'ambito in cui succede, c'è una sola cosa: la paura. la paura. Da una parte, la paura di morire o di non essere curati e, dall'altra parte, la paura di non poter curare come vorremmo e potremmo da medici.

E la paura blocca: blocca la mente, il cuore e fa tremare le mani, quelle mani che fanno sì che tu sia un buon medico. Queste sono le parole che provengono da alcuni sanitari commentando questo disegno di legge.

Grazie si trova di fronte un paziente che vede come sua potenziale controparte, un potenziale attore in un procedimento civile che chiede il risarcimento dei danni e che denuncia davanti alla procura,

il paziente, nel momento in cui entra in una struttura e si mette nelle mani di un medico, prima va dall'avvocato per vedere come riuscire a trovare delle soluzioni per un domani. Non dobbiamo agire per prevenire una eventuale causa; dobbiamo cercare di costruire il più possibile un clima di assoluta collaborazione. Ripetiamo, medico e paziente sono dalla stessa parte.

Ogni qualvolta nasce un bambino, si è di fronte a una delle più grandi responsabilità. Un neurochirurgo che interviene all'interno del cranio e opera su superfici minime, si trova ad avere delle proposte di polizze per ipotesi di responsabilità elevatissime. Ma non siamo in quei Paesi stranieri dove i medici guadagnano 150.000 euro all'anno. Stiamo parlando di medici, che operano nelle nostre strutture prendendosi delle responsabilità enormi, che non arrivano a 2.000 euro. È questa la cosa che non ha senso. Pertanto, ci auguriamo

Abbiamo visto come siano diminuiti i finanziamenti e la spesa per la sanità pubblica in questi anni. Una sanità, la nostra, che conta liste di attesa improponibili per un esame diagnostico, ritardi che foraggiano la corruzione e creano un doppio binario di pazienti: quelli che devono attendere a discapito della loro salute e quelli che hanno una corsia preferenziale, perché pagando riescono a sopperire alla mancanza. Oltre 200 procedure diagnostiche rese a pagamento, aumento dei *ticket* e sempre più persone che rinunciano al fattore prevenzione a causa degli elevati costi e delle suddette attese: mesi per una risonanza magnetica; un anno per una mammografia o una TAC. Capirete bene che viene a perdersi, ovvero a stravolgersi completamente il termine di diagnosi preventiva. Potrà effettivamente cautelarsi soltanto chi, a pagamento e privatamente, potrà saltare la fila. Vi rendete conto che tra ritardi e disorganizzazione dovuti a mancanza di risorse e finanziamenti, a una gestione spesso sconsiderata da parte dei dirigenti che gestiscono gli ospedali, la gente si vede costretta a rinunciare alle cure? Questo sarebbe il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione? Lo dimostrano i dati, perché è in costante aumento la spesa sanitaria annuale sostenuta dai pazienti di tasca propria. e prima e meglio ti curi. Dopo di che cosa importa della stragrande maggioranza della popolazione che già a stento riesce ad arrivare alla fine del mese? Bella uguaglianza, onorevoli colleghi! A me sembra che con questo disegno di legge si cerchi di voler mettere le mani avanti, se consideriamo anche la situazione in cui versa il personale sanitario. Infatti, nella stragrande maggioranza dei nostri ospedali si assiste ad una grave carenza di personale e l'età media dei lavoratori è sempre più alta a causa della mancanza di *turnover*. Tutte le ore mancanti non vengono mai coperte, se non a discapito del personale rimasto in servizio con turni massacranti, sottopagato poi rispetto agli altri colleghi europei. Sono in aumento, tra l'altro, a causa delle situazioni di sofferenza, i casi di sindrome da *burnout*. Tutto ciò mentre sempre più giovani infermieri e ostetriche sono costretti a rifugiarsi in altri Stati europei per vedersi garantito un tenore di vita degno di questo nome. Nonostante questo marasma, che si traduce in carenza di diritti con cui si infrange la nostra Costituzione, che si fa? Invece di sanare la critica situazione attuale si va ad intaccare ancora maggiormente la posizione dei pazienti. Mentre fino a oggi era il medico a dover dimostrare che il danno provocato al proprio paziente non fosse la conseguenza della sua azione colposa, oggi è il paziente stesso a dover dimostrare l'esistenza del caso di malasanità avvenuto a suo discapito, che ricordiamo essere la parte debole in questo rapporto, colui che non potrebbe mai avere gli strumenti tecnico-scientifici e le conoscenze adeguate per comprendere la portata dell'errore o negligenza di un medico; lo stesso che dovrebbe procurarsi informazioni da quelle stesse strutture coinvolte che naturalmente non avrebbero alcun interesse a collaborare effettivamente e che si sa potrebbero sempre tirare fuori cartelle vaghe e imprecise. Quindi, caro paziente, avrai liste di attesa lunghissime, molto spesso dovrai pagare di tasca tua, ma se e quando riuscirai a curarti e si verificherà un danno a tuo discapito sarai tu stesso, vittima, a dover dimostrare la negligenza e l'impreparazione del dottore. Senza contare che si parla di un fantomatico fondo senza avere nessun'altra certezza a riguardo. Verrà esclusa la responsabilità penale del medico, anche per colpa grave, se se rispetterà le buone pratiche e le linee guida previste, come a dire che ci si potrà trincerare al sicuro dietro un testo, evitando l'adozione delle scelte terapeutiche più

con il loro operato, ma salvi dalle linee guida, continueranno ad operare nelle stesse strutture mettendo in pericolo altri pazienti. Forti dubbi mi suscita, poi, l'effettivo ruolo delle società scientifiche in quanto unici soggetti legittimati a produrre le linee guida considerando, soprattutto, Grazie più che altro, su come si gestisce la sanità pubblica e gli ospedali per favorire davvero i pazienti, assicurare una effettiva uguaglianza e non intercedere sempre e solo a favore delle potenti *lobby*, promettendo finanziamenti e posti di lavoro solo per fini propagandistici. Pertanto, nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, annuncio il mio voto contrario. Signora Presidente, onorevoli colleghi, ormai da molto tempo si è diffuso nell'opinione pubblica un senso di diffidenza nei confronti degli operatori sanitari, nell'errata convinzione - come è stato detto da qualche altro collega - che la medicina sia onnipotente, una scienza esatta, cosa che non è: come è stato detto, la medicina è un'arte praticata da uomini nei confronti di altri uomini. Un eventuale risultato sfavorevole è sempre stato quindi letto dal paziente come riconducibile ad un loro inappropriato comportamento o ad una inadeguatezza del funzionamento delle strutture assistenziali. I dati a nostra disposizione ci dicono che dal 1994 al 2015 il numero dei sinistri da responsabilità professionale medica denunciati si è triplicato, arrivando arrivando fino a 34.000 casi. Vi è stato quindi un aumento delle denunce sia nei confronti di singoli medici, sia nei confronti delle strutture sanitarie (circa 20.000) con un aumento del 255 per cento rispetto al 1994. tutto ciò sia anche legato ad una cattiva informazione da parte degli organi di stampa, che spesso preferiscono fare sensazionalismo, perché fa molta più *audience*

lo *scoop* ed il sensazionalismo. Tutto questo ingenera la paura e la diffidenza dei cittadini nei confronti della sanità italiana, che tra l'altro è una delle migliori al mondo, e dei medici italiani, che pure sono fra i migliori al mondo.

che è centrale nell'impianto del provvedimento, è stato integralmente sostituito a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 6.100. Possiamo quindi dire che complessivamente si è fatto un buon lavoro. Oltre alla riformulazione dell'articolo 6, vorrei ricordare brevemente i contenuti più interessanti di questo provvedimento. All'articolo 2 si prevede, per esempio, che le Regioni possano affidare all'ufficio del difensore civico la funzione di garante del diritto alla salute. In ogni Regione è istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, con la funzione di raccogliere i dati sui rischi e gli eventi avversi al contenzioso generato e di trasmetterli all'Osservatorio nazionale per le Buone Pratiche sulla sicurezza della sanità, che poi provvederà ad individuare le idonee misure alla prevenzione e alla gestione del rischio sanitario. Questo è molto importante: si fa cioè una sorta di prevenzione dei rischi, perché raccogliendo tutta la casistica si può vedere dove ci sono

Sulla trasparenza dei dati viene previsto che la direzione sanitaria della struttura sanitaria, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, fornisca la documentazione. Questo è volto certamente alla tutela e alla maggiore trasparenza nei confronti del paziente. All'articolo 8 viene inserito il tentativo obbligatorio di conciliazione con l'obbligatorietà di partecipazione non solo di tutte le parti, ma anche delle compagnie di assicurazione, che sono soggetto importante, com'è emerso nel dibattito in Assemblea su questo aspetto, che bisognerà ulteriormente monitorare e su cui Pensiamo che questo possa essere uno strumento efficace per prevenire la proliferazione dei contenziosi, che come al solito ingolfano anche le aule giudiziarie. Non è inutile infatti ricordare, cari colleghi, che il 95 per cento dei procedimenti penali per lesioni personali colpose a carico di esercenti della professione sanitaria si conclude si conclude con un proscioglimento mentre, per quanto riguarda la sede civile, le richieste di risarcimento vengono accolte solamente nel 34 per cento dei casi. Questo la dice lunga sulla giustezza

Grazie agli eventi accaduti nei dieci anni precedenti alla conclusione del contratto assicurativo, anche se si sarebbe potuto specificare meglio in ordine ai contenuti della polizza assicurativa e all'operabilità temporale della medesima.

nel formulare l'articolo 15 riguardante la nomina dei consulenti tecnici e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Rimane ferma infatti la necessità che in questo tipo di giudizio, proprio per la sua delicatezza, sia necessario che i consulenti e i periti nominati abbiano cognizione di causa della materia. Ecco perché avevamo ritenuto che l'individuazione e il coinvolgimento, per esempio, delle società scientifiche che hanno redatto le linee guida sarebbe stato assolutamente positivo.

Da taluni questo provvedimento è stato salutato come un risultato storico. Noi, molto più prudentemente, pensiamo si tratterà di una buona legge, di un buon inizio che poi, come tutte le leggi fatte dagli uomini,

D'altra parte, il tema biopolitico è molto dibattuto già dalla sua iniziale definizione di Michel Foucault che la definisce una sorta di dominio della vita, declinata attraverso un dominio della politica sulla vita e della vita stessa. Qualcuno mi potrebbe chiedere perché questo tipo di argomentazione; noi non possiamo esprimere un giudizio in merito ad una legge, non possiamo esprimere un parere favorevole o no, se non analizziamo il contesto culturale, i principi e i valori di riferimento. A me preme sottolineare qual è lo stato attuale - lo dico da clinico, da senatore e da bioeticista - per quanto riguarda il riduzionismo sociale che caratterizza non la relazione - attenzione ai termini in ambito bioetico e biopolitico - ma il rapporto medico-paziente. Questo perché il rapporto medico-paziente è un'anonimia tra due soggetti che contrattualizzano la loro non relazione. Vale a dire che nella dimensione del sociale umano il riduzionismo si ricollega all'essere individuo che contrattualizza, medico con paziente, un comportamento assistenziale che possa essere il migliore possibile. Noi abbiamo dimenticato che nella dimensione del sociale umano

dell'attività assistenziale si chiama alleanza terapeutica, alleanza di cura, relazione medico-paziente. A me non sembra un rapporto, ma piuttosto una relazione che si basa su di un'alleanza che, ancor più che terapeutica, è un'alleanza di cura. Scusate, molte volte si usa questa sorta di sinonimia tra cura e terapia; eppure non è così: la terapia è infatti inclusa nella cura, ma non rappresenta la cura stessa. Vorrei richiamare alla vostra attenzione su una differenza sostanziale tra cura e terapia; la terapia non è altro che un evento che si realizza nella contingenza di uno stato patologico; quindi, usando una terminologia propria nell'ambito della filosofia e della bioetica, una realtà di ordine ontico. Ne viene di conseguenza che la relazione nasce nella contingenza di una patologia. Non può essere però la terapia sinonimo di cura, perché la dimensione della cura, che è propria anche della realtà non solo assistenziale medica, ma anche socio assistenziale, è la dimensione ontologica di due persone che si incontrano in una riconosciuta fragilità. Ed è quella fragilità di essere umano in quanto paziente che trova nell'altro, in quanto medico, il suo alleato. Credo che ciò rappresenti la finalità di questo disegno di legge, una finalità che si è cercato di tradurre in norme che, anche se non perfette, in quanto perfettibili iscritte nelle cose della natura umana, pur tuttavia cerca di ricomporre quel rapporto e ritradurlo in una dimensione di relazione. Ma per quale motivo? Perché già di per sé è difficile dar luogo ad una relazione tra due soggetti quando vi è una diversità di ordine antropologico, di ordine contenutistico e direi ancor più di ordine semantico. Noi sappiamo come esista un vero e proprio conflitto nel rapporto medico-paziente, un conflitto tra principi fondativi, tra libertà e bene e tra che cosa si intenda per libertà da parte del medico e come questa, invece, venga declinata dal paziente stesso, e che cosa rappresenti il bene, se rappresenta il bene totale della persona in quanto paziente oppure un bene semplicemente meccanicistico o di ordine biomedico. Inoltre, l'altro conflitto è tra autonomia e beneficità: su questo vorrei soffermarmi qualche secondo per un motivo molto semplice, perché nell'ambito del rapporto medico-paziente è sempre la declinazione dei quattro principi del cosiddetto principialismo anglosassone di Beauchamp e Childress. Per costoro sono quattro i principi che uniformano il rapporto medico-paziente: il principio di giustizia, il principio di autonomia, il principio di beneficialità e il principio di non maleficenza. Se dovessimo porre questi quattro principi sullo stesso piano, non riusciremmo a trovare davvero un principio assoluto di riferimento che possa prevalere sugli altri. Eppure tra

stessa. Il senatore Laniece ha presentato un disegno di legge in merito, dando luogo quindi ad un miglioramento attraverso la telemedicina introdotta in un disegno di legge, non solo all'assistenza sanitaria ma anche alla fruibilità delle cure e alla diagnosi precoce. Certo, non sono mancate alcune osservazioni critiche poste da alcuni in merito al disegno di legge stesso. Una di queste vorrei sottoporla alla nostra attenzione

Ne viene di conseguenza che attraverso la rideclinazione corretta del consenso informato, di cui devo dire questo provvedimento aveva assolutamente bisogno ma che è stato rimandato ad altro progetto di legge in corso di esame

sul consenso informato si arrivi a una puntualizzazione che sia estremamente dettagliata perché solo così, attraverso un consenso

non solo dei medici, ma di tutti coloro che sono coinvolti per il bene e la salute del paziente. Credo che questo possa rappresentare un aspetto importante del disegno di legge, che cerca di riproporre un'alleanza attraverso una ridefinizione per quanto riguarda la responsabilità civile e penale, in modo da ridurre quella deriva che caratterizza proprio la medicina difensiva oggi è ampiamente e massivamente presente sia nella formulazione della medicina difensiva positiva

si è cercato di fare in modo che dalla dimensione di "stranieri morali", propria del contrattualismo, si passasse all'espressione "amicizia morale". Dal solo principio di autonomia, che caratterizza oggi il contrattualismo, si cerca di passare alla beneficità,

dalla separatezza che caratterizza, ancora una volta, il contrattualismo alla relazione del noi, che caratterizza invece il personalismo;

finestra"). Le nostre tribune oggi sono molto affollate e, quindi, dobbiamo fare un certo numero di saluti. Sono presenti gli allievi e i docenti del Liceo scientifico «Antonio Gallotta» di Eboli, in provincia di Salerno, che stanno nel primo ordine delle nostre tribune.

Sinistra Italiana conferma il voto contrario al disegno di legge che avrebbe dovuto avere l'obiettivo importante di offrire un quadro giuridico più chiaro e di maggior tutela per gli operatori sanitari e di provare a semplificare il contenzioso medico-paziente. In realtà, oggi ci troviamo dinanzi a un disegno di legge che garantisce una maggiore tutela giuridica ai professionisti sanitari, alle aziende sanitarie sia pubbliche che private, rispetto all'azione del risarcimento di danni, ma non c'è un uguale aumento delle garanzie e delle tutele per i cittadini pazienti. Si sarebbe potuto fare molto di più per bilanciare il diritto dei cittadini e delle cittadine di vedere riconosciuto il torto e il danno subito e, contestualmente, garantire una maggiore tutela ai medici e al personale sanitario, pur nell'autonomia dell'esercizio della professione. La libertà di azione del medico risulta invece limitata perché vincolata a precise linee guida, che diventeranno non più strumenti facoltativi di consultazione e di riferimento, bensì strumenti che rischieranno di imprigionare l'autonomia del medico e fondamentali per la tutela della responsabilità. Si scarica sul malato l'onere della prova di un'eventuale malasanità, malato costretto a districarsi tra natura contrattuale ed extracontrattuale della responsabilità; e tutto diventerà più complicato in un settore già di per sé di difficile interpretazione e accertamento. Ma forse questo è proprio l'obiettivo che si voleva perseguire: ci sarà anche quella che si chiama giuridicamente l'inversione dell'onere della prova. Insomma il cittadino, per far fronte a questo nuovo onere, dovrebbe avere conoscenze scientifiche e della dinamica degli eventi che ovviamente non ha, dovrebbe avere accesso a informazioni che non sono sempre nella sua disponibilità, dovrebbe avere a disposizione prove, chiedendole a chi ha più poteri di lui e non ha alcun interesse a dargliele e che farà di tutto per ostacolare anche gli obblighi sulla trasparenza. Insomma, come fa materialmente un malato a provare la responsabilità del medico nelle migliaia e migliaia di casi clinici diversi, diversi, con tutte le loro infinite complessità? Si sarebbe potuto fare di più per riequilibrare il diritto dei cittadini a vedere riconosciuto il torto subito e, contestualmente, per garantire una maggiore serenità ai medici e al personale sanitario; ma questo equilibrio non è stato rispettato. Siamo infatti dinanzi a una evidente diminuzione del livello di tutela del cittadino vittima di sanità. Si pone una limitazione per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, circoscrivendo la responsabilità degli operatori sanitari alle sole ipotesi di colpa grave ed escludendo addirittura dalla nozione di colpa grave le ipotesi in cui, fatte salve le rilevanti specificità del caso concreto, siano state rispettate le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge. È evidente che questa limitazione restringe in modo rilevante l'ambito di tutela di chi usufruisce della prestazione sanitaria e ciò si rileva ancora più grave nel sistema penale, che pone al centro di tutto il sistema di accertamento e repressione dei reati il valore della vita e dell'incolumità fisica. Questo era già tutto accaduto con il decreto Balduzzi e con i tre anni di applicazione, che avevano ben evidenziato tutto questo. Sulla limitazione della responsabilità penale alla sola imperizia, con esclusione della negligenza e dell'imprudenza, parametri necessari per definire la colpa penale (come tanti colleghi hanno spiegato anche oggi, nei loro interventi, e nei mesi precedenti, in cui abbiamo affrontato la discussione di questo disegno di legge), la Corte di cassazione si è già divisa, lasciando intendere le problematicità e le falle di questa limitazione. Oggi, con questo disegno di legge, ci portiamo dietro e consolidiamo ulteriormente le storture che avevamo evidenziato in tanti nel decreto Balduzzi. Nel testo è stata tolta una parte importante, quella che riguardava il rischio clinico, tutte norme di prevenzione e gestione del rischio sanitario che avrebbero potuto far sì che tutte le strutture, pubbliche e private, attivassero una funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario. Tenere insieme il rischio clinico e la responsabilità avrebbe avuto un valore diverso. Nel provvedimento c'è un tema delicato, che riguarda il sistema delle assicurazioni e la scelta di molte Regioni, in questi anni, di smettere di pagare le assicurazioni delle aziende e dei medici che avrebbero potuto tutelare anche i professionisti e non solo le Questo ha aperto ad un vero mercato assicurativo e comprendiamo bene la necessità di inserire almeno i minimi sui premi assicurativi; ma si è deciso di abbandonare i cittadini e il sacrosanto diritto alla tutela della propria incolumità, esponendoli a molte incertezze e lungaggini giudiziarie e burocratiche. burocratiche. E siccome spesso parliamo di danni subiti nel momento in cui invece si cerca aiuto per la propria salute, ci saremmo aspettati un sistema che si carico, al di là delle truffe, del cittadino in difficoltà e non un sistema che si difende. Questo è particolarmente grave quando si parla di strutture pubbliche. Insomma, per noi ci sono criticità, tante questioni aperte e una certezza: la legge rappresenta uno scambio tra la tutela, l'impunità giuridica e l'autonomia del medico e indebolisce la tutela dei diritti dei cittadini. Siccome sono in gioco interessi costituzionalmente rilevanti, come il diritto alla salute, non può bastare una strozzatura delle vie d'accesso alla giustizia senza indagare le vere ragioni della malasanità, che è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale, legato troppo spesso a tagli e a scelte politiche sbagliate, come nell'ultimo caso di cui tutti hanno parlato. Mi riferisco alla vicenda di Nola, che in questi giorni è sui giornali, dove si fa finta che non esistano gravi responsabilità politiche di chi governa la sanità in quella Regione. Forse sarebbe stato maggiormente necessario intervenire anche sui tempi della giustizia, perché questo è uno dei temi che riguardano la possibilità di tutela dei cittadini. Vorrei infine aggiungere, tra le criticità

vorrei ringraziare il relatore, la Commissione sanità e l'Assemblea nella sua interezza, naturalmente nel rispetto delle diversità che sono emerse anche in sede di dichiarazione di voto. Riteniamo, però, doveroso da parte nostra fare ancora qualche breve e ulteriore precisazione proprio per rafforzare

a precisare un aspetto fondamentale: noi riteniamo che il rapporto tra medico e paziente non sia un'alleanza; lo gridiamo con forza, signora Presidente. È un rapporto basato sulla fiducia tra due soggetti, per cui il medico o l'operatore sanitario,

due, ma sono gli aspetti fondamentali per cui un medico o un operatore sanitario deve rispondere alla richiesta di qualità di prestazione, alla richiesta di salute: la scienza e la coscienza. Non ci sono altri riverberi; non può esserci alcun tentennamento o *escamotage* giuridico, pur nel rispetto dei colleghi che hanno fatto valutazioni squisitamente giuridiche, circa l'approvazione di questa norma. Riteniamo che la competenza era e rimane della Commissione sanità, sanità, proprio in virtù del fatto che si tratta di rapporto tra medico e paziente/utente, di una richiesta di salute,

buone prassi, che è di garanzia non solo per il medico, ma anche per il paziente. Ci sono infatti momenti in cui il medico si trova nella necessità di ragionare scientificamente con la propria coscienza e che avere la possibilità di ritenere che l'adeguamento alle linee guida non è un atto di scienza,

volte ad un'ulteriore umanizzazione del rapporto. Su questo tema saremo sempre pronti a intervenire e collaborare. Quello che ci preme è soprattutto garantire sempre di più che questo rapporto sia lineare e basato sulla

come frutto della necessità di regolare il contenzioso tra controparti. In nessun passaggio il provvedimento sottolinea e garantisce quello che dovrebbe essere lo spirito ispiratore di una legge a tutela delle migliori cure possibili, cioè che il paziente cittadino e l'esercente la professione sanitaria non possono essere visti come controparti, posto che solo un rapporto di fiducia reciproca, nel contesto di regole a tutela di entrambi, può essere la base su cui edificare un'assistenza sanitaria giusta e di qualità elevata per chiunque e in qualsiasi situazione. Nonostante l'articolo 1 sancisca che la sicurezza delle cure sanitarie sia una parte costitutiva del diritto alla salute e metta in campo misure per la gestione del rischio clinico, appare non del tutto sufficiente quando non si attuino le condizioni perché ci sia un rapporto paziente e personale sanitario: infatti, da professionista più che per il *risk manegment* aziendale avrei preferito che la tempistica per un agoaspirato ecoguidato della tiroide che debbo fare non fosse di soli 12 minuti.

Riconosco al relatore un grande sforzo di sintesi e di mediazione, ma cercare un equilibrio tra i diversi interessi non è stato sempre possibile; ritengo tuttavia che in diversi ambiti il compromesso raggiunto sia accettabile ed in alcuni passaggi, come l'articolo 16, sicuramente pregevole.

alcuni punti non ci convincono del tutto, soprattutto dal punto di vista della responsabilità professionale, in quanto l'articolo 6 contiene una previsione peggiorativa rispetto alla disciplina attuale (legge Balduzzi). Inoltre, anche sul piano civile abbiamo l'impressione che alcune norme siano potenzialmente lesive del principio di uguaglianza e parità in giudizio e del contraddittorio tra le parti.

in quanto abbiamo visto che c'è una fortissima asimmetria tra il mondo assicurativo e le professioni sanitarie a svantaggio di queste ultime e di conseguenza anche dei pazienti. Inoltre, anche mutuare alcune valutazioni

uffici legali in maniera più chiara nell'aiuto ai professionisti, anche perché questo è stato un problema che ho vissuto personalmente e quindi da questo punto di vista capisco quando sia complicato.

Queste figure professionali indispensabili sono fortemente tutelate in questo articolo e per questo dovrebbero essere particolarmente attenti all'etica ed alla correttezza del loro lavoro,

fanno partire contenziosi a danno non solo del paziente, ma della struttura sanitaria e del professionista, che terminano poi in nulla, contando su un sistema che rarissimamente li vede poi valutati. Forse Forse sarebbe stato opportuno considerare anche questi comportamenti come aggravanti e forse in questo caso speriamo che gli ordini professionali possano intervenire, quanto meno in un ambito Per le ragioni sopra esposte, seppur riconoscendo che il testo presenta elementi di maggior equità rispetto a quello approvato dalla Camera, annuncio il voto di astensione del Gruppo Movimento 5 Stelle.

stante anche la situazione storica che si è sviluppata in ambito sanitario, avesse una certa urgenza. Mi riallaccio a quanto detto dalla collega del Gruppo SEL relativamente al fatto che i componenti della Commissione sanità non abbiano bene accolto la modalità di gestione dell'Aula relativamente a questo provvedimento, visto e considerato che, spesso e volentieri, purtroppo, il precedente Governo dava indicazioni con innumerevoli decreti-legge, per cui l'emergenza superava sempre l'ordinarietà. Questo va rimarcato. Sottolineo anche io, come hanno fatto altri colleghi, la positività dell'azione svolta e della discussione in Commissione sanità su questo provvedimento.

è dovuto al lavoro di tutti i commissari, in assoluto. Il provvedimento richiedeva una certa urgenza, perché è fuor di dubbio, soprattutto anche per responsabilità della parte mediatica in generale,

sanità. Detto questo dal punto di vista generale, il provvedimento presenta degli aspetti molto positivi, ma anche delle luci ed ombre, secondo la mia personale opinione. Nel senso che non vorrei

la sanità non funziona. E qui sorge anche un problema di giustizia e di tempistica, perché il provvedimento agisce nel merito, ma quando poi la giustizia impiega anni e anni per dare un riscontro in un senso o nell'altro anche questa è una colpevolezza dello Stato nel merito. Il provvedimento, secondo me, ha cercato di trovare un giusto equilibrio tra le responsabilità del medico, quindi le garanzie per quanto riguarda il personale sanitario, e la possibilità da parte del cittadino di rivalersi quando subisce della malasanità. E questo è estremamente importante. C'è poi il capitolo delle assicurazioni, che veniva prima ricordato dalla Presidente della Commissione sanità per quanto riguarda il problema della concorrenza, perché è non sostenibile il fatto che veniva ricordato, ossia che ci siano delle società di assicurazioni che non siano disponibili e che si facciano dei cartelli per cui la polizza abbia dei costi assolutamente inaccessibili sia per il personale medico che per le strutture. Mi auguro che le tempistiche per le linee guida e per questo aspetto più squisitamente burocratico trovino sostanzialmente

e sanitario diventa un elemento fondamentale. Bene ha fatto, secondo me, il Parlamento ad occuparsene, malgrado ci siano, come detto prima, alcune zone d'ombra e alcune caratteristiche che devono essere migliorate,

è stato proprio quello sulla responsabilità professionale, allora chiamata rischio clinico o responsabilità del medico. È passato un certo numero di anni ed arriviamo oggi ad un'approvazione che io trovo straordinaria. Capisco che non sempre siamo stati chiari con i colleghi, e me ne scuso, ma il tema

non è vero, perché questo è un provvedimento che si colloca al centro non di una manutenzione del sistema sanitario, ma di una vera e propria strategia di riforma. Questo provvedimento, accanto a quello sul riconoscimento delle professioni sanitarie e sulla riforma degli ordini (che - voglio ricordare - il Senato ha licenziato e che ora è alla Camera e mi auguro che lo approvi rapidamente), sono due capisaldi, anche perché in Italia mancavano completamente leggi in materia. Noi parliamo dell'Europa, di medicina transfrontaliera, della possibilità di cura in tutta Europa, di qualità europea dei servizi sanitari, ma l'Italia era indietro: l'Italia non era in Europa Europa e non vi è ancora finché non saranno approvate queste leggi che sono norma comune in larghissima parte dei Paesi dell'Unione europea. È stato detto molto sul merito del provvedimento. Mi permetto però di dire

quanto è stato affermato in quest'Aula e cioè che, in realtà, il provvedimento ha subìto un rallentamento nei lavori dell'Aula per problemi politici sul provvedimento medesimo. Non è così; lo dimostra il clima che c'è stato in Commissione, un clima ampiamente positivo,

Vengo ad alcune considerazioni molto brevi: partiamo innanzitutto dal riconoscimento che è giunto da parte delle associazioni dei pazienti del miglioramento del disegno di legge nel lavoro che abbiamo svolto al Senato. È molto importante perché segnala la dignità del cittadino accanto alla dignità del professionista della sanità. Credo che questo sia un riconoscimento un riconoscimento importante per il valore del Servizio sanitario nazionale, perché si è parlato di alleanza tra medico e paziente. Dico di più: con questo provvedimento passiamo da un approccio individuale al problema della responsabilità a un approccio partecipativo e a un coinvolgimento più attivo del paziente. La possibilità di richiedere la cartella clinica è certamente una sfida per un intero sistema, perché

e il diritto del personale sanitario nel suo complesso, a partire dal mondo medico. Le norme servono a rendere dinamico un sistema. A chi dice che, in realtà, è un provvedimento insufficiente dico invece che è un provvedimento che mette le basi perché si possa lavorare in modo diverso e organizzare il sistema in maniera diversa, a cominciare che pone l'assicurazione a carico della struttura, tema importantissimo che richiede un rapporto, anche con il mondo assicurativo, con il mondo assicurativo, davvero differente rispetto al passato. Ma di questo abbiamo già ampiamente trattato. Il terzo punto di grande rilievo è quello che riguarda la ricerca e la presa in carico da parte dell'Istituto superiore di sanità dell'accreditamento delle linee guida. Badate che è un punto non irrilevante, perché finalmente c'è un ente di riferimento certo e controllato dal Ministero della salute per tutto ciò che riguarda la ricerca e l'evoluzione della ricerca clinica e una maggiore sicurezza, quindi, con una validazione ufficiale delle scelte che vengono compiute quotidianamente nei confronti della persona che ha bisogno di assistenza. Si tratta di un tema che ha davvero al centro la dignità

dell'evento avverso. Non vorrei mai più vedere le pubblicità che abbiamo visto in televisione, con quel microfono che diceva in modo così volgare: «Hai un problema sanitario? Ti hanno fatto del male? Rivolgiti a noi». Noi sappiamo che le cause nel campo della sanità solo il 2 per cento di queste centra l'obiettivo. Quello che però non si può tollerare è l'utilizzo del dolore e della malattia per fini di carattere commerciale. Questo riguarderà anche le assicurazioni, certamente riguarda anche le assicurazioni: il versante professionale in questi anni ha vissuto momenti drammatici. Siamo arrivati ad un punto in cui per un giovane medico pagare 10.000 o 11.000 euro di assicurazione annua significava di fatto non poter lavorare. non poter lavorare. E ancora, sempre nel campo delle assicurazioni, c'è stata una fase in cui nessuna società voleva più assicurare perché non c'era più credibilità. Con questo disegno di legge questa credibilità ritorna, perché si pongono pongono le premesse non soltanto di una solvibilità, ma anche della necessità di regole chiare e trasparenti che non sfruttino per motivi di mercato la dignità professionale né la dignità Grazie a tutti

a mio avviso segnala un'idea di riformismo nuovo, di riformismo vero, circa la possibilità di non cercare sempre la testimonianza, di non cercare di andare sempre

Io rispondo che ce l'abbiamo fatta, e non rispondo solo a quelle 5.000 persone, ma a tutti gli italiani ed alle italiane, alle persone che vivono sul nostro territorio che oggi c'è una possibilità in più una possibilità in più per il diritto alla cura, per quella cultura della sicurezza che è a tutto tondo e che pervade e deve continuare ad essere presente nel lavoro quotidiano del Servizio sanitario nazionale,

essere un nemico del bene, ma la perfezione è sicuramente un nemico mortale di entrambi». Sappiamo che siamo imperfetti, ma sappiamo che oggi abbiamo scritto una piccola pagina per il diritto alla salute.

vorrei ringraziare lei e tutti i Presidenti che hanno in queste settimane guidato i lavori d'Aula, la discussione e il voto sul provvedimento. Volevo ringraziare tutti i componenti dell'Assemblea, indipendentemente dalle loro appartenenze; li ringrazio per aver testimoniato la loro identità e la loro diversità, che assolutamente rispetto e che è preziosa per me e la mia cultura. Ringrazio i Ministeri e i Ministri coinvolti a vario titolo nel provvedimento: la ministra Lorenzin, il ministro della giustizia Orlando, i Sottosegretari che hanno presenziato ai lavori d'Aula e di Commissione, il sottosegretario Faraone, cui rivolgo sinceri auguri. Volevo ringraziare anche tutti i componenti della 12a Commissione, la Commissione referente del provvedimento, ed in particolare la presidente De Biasi. L'avete ascoltata e avete capito anche quanto sia stata preziosa ed indispensabile la sua guida nel portare in porto un provvedimento così complesso. In questo contesto ringrazio anche il consigliere Biancolatte e tutto l'Ufficio della Commissione per il preziosissimo lavoro svolto. Grazie dunque a tutti; grazie per il lavoro fatto. Come già detto dalla presidente De Biasi, la perfezione non ci appartiene, ma insieme - e di questo ne sono felice - abbiamo lavorato per un buon provvedimento.

La seduta è tolta